L'esame del decreto-legge in materia economico-fìnanziaria, per il quale sono stati ampliati i tempi già ripartiti tra i Gruppi, si concluderà nella seduta pomeridiana di domani. Domani mattina, alle ore 12,45, saranno poste ai voti le dimissioni presentate dal senatore Bettini. Anche per il decreto-legge in materia di pubblica sicurezza, che inizierà a conclusione del decreto finanziario, si è proceduto ad una nuova ripartizione dei tempi tra i Gruppi. calendario della prossima settimana, oltre ai provvedimenti già previsti (eventuale seguito del decreto-legge sicurezza, collegato servizi pubblici locali e ratifiche di accordi internazionali), reca anche il disegno di legge in materia di semplificazione di adempimenti amministrativi sanitari. Sono inoltre previste due sedute di *question time* con trasmissione diretta televisiva: giovedì 29 novembre, su questioni attinenti la RAI interverrà il Ministro delle comunicazioni; giovedì 6 dicembre, il Ministro per i rapporti con il Parlamento risponderà sui Comuni di confine e il Ministro dei trasporti su quesiti relativi al taglio di treni pendolari e a lunga percorrenza, al gruppo Tirrenia e all'aeroporto di Vicenza. sera chiuderemo i lavori alle ore 19 per dare un po' più di tempo alla Commissione affari costituzionali che sta discutendo il decreto sicurezza.

Onorevoli colleghi, il 24 novembre nella valle di Paghman, una località a circa 15 chilometri da Kabul, perdevano la vita a seguito di un attentato suicida il maresciallo capo dell'Esercito Daniele Paladini, del Secondo Reggimento Pontieri di Piacenza, e nove civili afghani, tra cui quattro bambini; altri tre militari italiani rimanevano feriti insieme a numerosi civili. Sono certo di interpretare il pensiero di tutta l'Assemblea ricordando in apertura dei nostri lavori tutte le vittime di questo atto inumano e il sacrificio di un uomo che, senza esitazione, a costo della sua vita ha operato per consentire l'individuazione dell'attentatore, riducendo così sensibilmente un ben più tragico possibile bilancio. Un atto di generosità, quello del maresciallo capo Paladini e di tutti i militari italiani, che incarna lo spirito della nostra missione in quella terra, come delle altre nostre missioni: spirito sempre proteso ad affermare la vita e la speranza in aree sfigurate dalla guerra e dalla violenza. I militari italiani si trovavano in quella zona per l'inaugurazione di un ponte che li aveva visti impegnati nella ricostruzione; un luogo scelto non a caso dall'attentatore per distruggere oltre la vita anche la possibilità di una rinascita civile e sociale di un Paese già duramente provato. Il Senato della Repubblica si stringe attorno alla famiglia del maresciallo capo Paladini e alle famiglie delle vittime civili e ai militari italiani impegnati nelle missioni all'estero; ai militari italiani feriti auguriamo un pronto ristabilimento. Vi invito ad osservare un momento di raccoglimento.

volevo informare il Senato di un fatto molto grave in sé e anche per il contesto in cui è avvenuto. Ieri notte, in un piccolo paese della provincia di Bologna, la signora Francesca Catalano, di 38 anni, è stata uccisa nella sua casa e e alla fine delle indagini il marito è stato arrestato. Questo fatto conferma la gravità, la rilevanza, la centralità assoluta del fenomeno della violenza contro le donne, del suo carattere pervasivo, costante e strutturale. Per essere più precisa e chiara, parliamo di "femminicidio", di questa guerra a bassa intensità contro le donne che semina non solamente morte, ma anche violenza, maltrattamenti e botte, anni abbiamo cercato di portare alla luce nello spazio pubblico della politica. Dobbiamo parlare di questo e non di altro. È una violenza di uomini contro le donne, che si annida prevalentemente nelle famiglie, nelle case. Nasce da antiche culture patriarcali che vengono alla luce, ma si mescola oggi anche alla rabbia distruttiva e nuova di uomini contro gli effetti della rivoluzione più lunga e più incruenta: quella delle donne. Tale questione dovrebbe essere argomento della politica e del Parlamento. Di questo dovrebbero parlare i giornali e non di altro, dichiarando il debito a quello straordinario movimento che ha riempito sabato le piazze e le vie di Roma e domenica le piazze d'Italia. Parliamo di questo e non di altro. Non rimuoviamo lo scandalo delle cause di questa violenza che troppo spesso la politica ha rimosso. La politica alta distingue ciò che è principale e ciò che è secondario: direbbero gli antichi filosofi, la sostanza dall'accidente. La manifestazione di sabato e il dibattito che l'ha preceduta questo ci chiede e ci dice di riflettere sulla violenza degli uomini contro le donne, che va fermata, sugli strumenti per fermarla nei luoghi in cui prevale, cioè nelle case; strumenti che non sono le politiche securitarie o le scorciatoie repressive, ma un impegno educativo e formativo e strategie sociali a sostegno delle donne.

accolti e condivisi dall'opposizione. Si è dovuto ricredere e non ha potuto presentarli per una questione che è stata poi discussa all'interno della Commissione

che anche il decreto-legge sulla sicurezza viene messo in discussione - e quindi arriverà probabilmente in Aula senza essere accompagnato dal relatore - per colpa dei talebani che sono all'interno di questa maggioranza.

Il tempo decorre dalla conoscenza. In questi giorni ho avuto conoscenza di un articolo intitolato «Notte della vergogna» nel quale, con riferimento alla seduta del Senato sul decreto fiscale, l'autore afferma che quella è una data della vergogna e che non bisogna «dimenticare le date della vergogna, persone, circostanze e situazioni che disonorano tutti». Non solo, ma parlando del Senato della Repubblica, signor Presidente, lo ha appellato come «uno dei locali peggio frequentati di Roma» e ancora, sempre con riferimento al Senato, lo ha considerato come «un luogo mal frequentato» e principalmente frequentato da teppisti teppisti impegnati «nel peggio, con il privilegio di non avere un'immagine da salvare». Credo, signor Presidente, che la tutela del Senato sia un suo problema.

dichiarando: «Cara signora, lei se l'è andata a cercare. Invece di stare al di sopra delle parti si è messa a votare. Dunque non si aspetti gli onori di casa». Come è facile verificare dalla comparazione con il resoconto stenografico, si tratta di un'affermazione assolutamente falsa. Ebbene, signor Presidente, al di là di questa falsità,

che, in più di un'occasione, è apparsa nelle cronache giudiziarie. Ho tolleranza per i comportamenti senili, anche quando sono furiosi e anche quando si correlano a presunzione e ad autoreferenzialità. Comunque, alla luce di questo articolo, mi si consenta di dire al senatore Colombo che ritengo sia una persona immeritevole di qualsivoglia considerazione e, in sintesi, un poveraccio!

nell'organizzazione dei lavori. Le ragioni della chiusura dei lavori sono quelle indicate dal collega Pirovano. Speriamo che i lavori dell'Aula portino ad una maggiore coesione, soprattutto nell'ambito del centro-sinistra.

Ritengo che la sacralità del Parlamento non consenta che colleghi scaglino l'uno contro l'altro accuse immeritate

Mi dispiace, ma non mi aspettavo dal senatore Nitto Palma un intervento di questo genere, che condanno totalmente. colleghi: il rispetto reciproco è una regola per tutti; ci tengo a ribadirlo fino in fondo e spero che questo invito venga rispettato

Presidente, qui vi è un falso, nel senso che l'ex ministro Castelli si riferisce ad un articolo nel quale difendevo Rita Levi-Montalcini dagli insulti ricevuti in quest'Aula. Invece, il povero Nitto Palma tentava di commentare il mio editoriale di domenica scorsa: sono due cose completamente diverse. Metterle insieme e citare estrapolando è un falso.

che non abbia un grande rispetto e una sensibilità forte per una donna che partecipa ai lavori quotidiani del Senato: quotidiani, non soltanto per i voti di fiducia.

il decreto ha subito alcune modifiche alla Camera, che è nostro dovere esaminare. lavoro della Commissione bilancio della Camera è stato finalizzato prevalentemente a intervenire su alcuni problemi legati alla copertura finanziaria delle norme uscite dall'esame di questo ramo del Parlamento. Si tratta di provvedimenti previsti, alcuni dei quali auspicati,

Si è posto rimedio a delle carenze nelle coperture finanziarie (alcune rilevanti) che avrebbero rappresentato un *vulnus* rispetto alle regole cui all'articolo 81 della Costituzione sull'adeguatezza, la congruità e la correttezza delle risorse destinate a finanziare gli interventi previsti; è inteso garantire la certezza che questi provvedimenti legislativi potessero essere adeguatamente attuati. Mi riferisco, in particolare,

in particolare in alcuni settori sociali più deboli, che non avrebbero potuto essere rispettate. Come dicevo, la correzione più rilevante è quella relativa agli incapienti, che riporta il *bonus* da 300 a 150 euro. L'emendamento approvato dal Senato aveva raddoppiato l'importo della detrazione e quindi anche quello della spesa, utilizzando come copertura finanziaria un fondo di 5 miliardi alimentato,

emotrasfusi e dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, vale a dire l'articolo 33 del testo al nostro esame. Tale norma prevedeva la copertura attraverso

n. 468. Considero la modifica apportata dalla Camera molto positiva, perché si è previsto di intervenire con una copertura più adatta

sull'aumento dell'accisa sui tabacchi sarebbe stata più adeguata a coprire una norma di carattere permanente.

è un vizio presente prevalentemente in alcuni settori sociali più deboli, il continuo aumento del costo delle sigarette può essere considerato non solo una tassa sul tabacco,

rispettivamente pari a 0,6 e 2 milioni di euro. Nel testo del maxiemendamento vi sono ulteriori modifiche in riferimento all'articolo 26,

al fine di non rinunciare ai fondi comunitari che, per essere acquisiti, necessitano di cofinanziamento. In particolare, viene introdotta una sospensione delle sanzioni a carico delle Regioni e delle Province autonome che non conseguono, nel 2007, l'obiettivo di spesa nel caso in cui lo scostamento registrato non sia superiore alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea e a condizione che lo stesso sia recuperato nel 2008. È una norma che ritengo positiva perché garantisce la possibilità di

con una diversa individuazione dei soggetti che dovranno essere i primi beneficiari, ovvero gli sfrattati e tra questi le giovani coppie, e non invece - come previsto originariamente - le giovani coppie e gli sfrattati. La modifica appare, ad avviso del relatore, opinabile, poiché nell'ambito della categoria degli sfrattati possono essere individuati soggetti altrettanto meritevoli dell'assegnazione di un alloggio, oltre alle giovani coppie. Infine, c'è la disposizione relativa

l'incremento delle detrazioni da 150 a 300 euro. Avevamo contestualmente approvato unacopertura finanziaria adeguata,

alle quali la copertura non avrebbe dato risposta sufficiente e concreta ed oggi non si creano più. Non concordiamo su questo. Riteniamo che

il decreto e quanto stabilito nel decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze, avranno diritto di beneficiare di questa detrazione, anche se

su una sentenza della Corte costituzionale che ha indicato dei punti fermi e dei vincoli in materia di decretazione d'urgenza che questo decreto-legge,

fino all'opinione pubblica, attraverso la trasmissione di questi dibattiti, le registrazioni e la lettura dei Resoconti. Questo decreto-legge vìola in pieno i punti fermi fissati dalla Corte costituzionale

politico-fattuale sulla situazione di emergenza e di straordinaria necessità che deve essere effettuata dal Governonel momento in cui ritiene di esercitare,

dell'80-90 per cento delle norme in esso contenute che nulla hanno a che fare con le infrastrutture, con il fisco, con gli incapienti.

che la Corte costituzionale ha deciso in maniera affrettata e non condivisibile, ma credo che sia innegabile che il decreto‑legge manca di un presupposto fondamentale. insegnato, o meglio dettato, un principio per cui anche il passaggio del decreto‑legge attraverso il Parlamento, Camera e Senato, non sana quel vizio originario. Vizio originario che riguarda

che non presentano quel sostegno dell'urgenza che deve avere il decreto-legge nel suo complesso o che sono estranee alle materie per le quali il decreto-legge è stato adottato dal Governo. Mi sembra un ragionamento semplice e lineare. Certamente può creare difficoltà nel governo della cosa pubblica

È evidente, infatti, che così facendo costringeremmo la Corte costituzionale, come è avvenuto per altre materie, dopo tanti buffetti e dopo il primo scapaccione, che è stato dato con l'ultima sentenza del 2007, ad usare il pugno di ferro anche per affermare un principio di autorevolezza della Corte stessa,

il relatore, senatore Ripamonti, ha esposto con grande precisione e completezza le poche modifiche che la Camera dei deputati ha apportato al decreto che stiamo esaminando.

le modifiche in tema di edilizia pubblica e di destinazione degli alloggi costruiti con lo stanziamento, ritengo sia da condividere la riserva sul merito del cambiamento operato alla Camera, nel senso che il venire meno di un privilegio nei confronti delle giovani coppie, sostituito da una preferenza verso le coppie in genere, suscita qualche perplessità proprio in virtù del carattere che l'assegnazione della casa acquista per le coppie che stanno creando una famiglia. Per quanto riguarda l'aspetto quantitativamente più rilevante, cioè la modifica delle norme sugli incapienti,

un ascoltatore ha posto al giornalista che stava conducendo la trasmissione un quesito proprio sul tema degli incapienti, domandando se, nella determinazione della platea degli aventi diritto, si sarebbe o meno tenuto conto del reddito familiare.

ha risposto che non era informato sul punto specifico, ma che, in effetti, riteneva che si sarebbe tenuto conto del carico familiare, cosa che notoriamente non è vera. vera. L'episodio ci fa cogliere tre aspetti: in primo luogo, che c'è un'attenzione diffusa tra la gente nei confronti di questo istituto; in secondo luogo, che quello che abbiamo fatto, qui e alla Camera, purtroppo non è abbastanza noto;

la soluzione di modifica che era stata trovata in questa sede andava in una direzione diversa e non teneva conto del problema: Quindi, credo che bene abbia fatto la Camera a a ritornare al testo originario, anche per gli aspetti tecnici di procedura su cui ha riferito il senatore Ripamonti. Vengo all'ultimo punto, che riguarda riguarda il Patto di stabilità regionale. Il senatore Ripamonti ha esposto le tecnicalità della questione, che hanno suscitato molte discussioni in Commissione bilancio;

Ciò di per sé non vuol dire che la disposizione sia buona, ma certo fa riflettere. In conclusione, vorrei sottolineare il carattere anche congiunturale della norma:

Si potrà discutere sull'efficacia di questo provvedimento di carattere congiunturale, ma certamente non si può negare la tempestività di fronte ad un peggioramento della situazione congiunturale: mi sembra, questo, un intervento opportuno. Del resto, tutto il decreto ha il carattere di un intervento congiunturale che ci fa sperare che la crisi economica, determinata dalla situazione americana, non colpisca il nostro Paese

torna oggi al Senato per essere definitivamente convertito in legge, dopo che la lettura della Camera ha introdotto modifiche ad otto articoli. Non si tratta di modifiche significative, se si escludono quella dell'articolo 44, che norma la misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito, e quella all'articolo 7-*bis*, che riguarda il Patto di stabilità delle Regioni. Ciò significa che il Senato della Repubblica in prima lettura ha lavorato bene, in modo ponderato, qualificato; nella sostanza, in modo efficace. Questo giudizio esce rafforzato se si considera la rilevanza economico‑finanziaria del disegno di legge per l'anno in corso. In effetti, la copertura riguarda una cifra considerevole: 8.407 milioni di euro. Siamo, in effetti, di fronte - è utile ribadirlo - al primo corposo atto della manovra economico-finanziaria 2007-2008 e in questo primo corposo atto vi sono misure di rilevante profilo sociale: il rifinanziamento degli asili nido, un programma straordinario per l'edilizia pubblica, fondi per la cooperazione internazionale, le disposizioni in favore di soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti, l'estensione dei benefìci riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, l'aumento di 150 milioni di euro per l'anno 2007 dell'autorizzazione di spesa per il 5 per mille, la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili, il potenziamento di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica per l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione e la realizzazione di immobili ad uso abitativo. Questo per ciò che concerne il sociale. [**Presidenza una migliore regolamentazione dell'uso delle biomasse; in particolare, i controlli introdotti sulla cosiddetta filiera corta e la moratoria di un anno dei processi di privatizzazione dell'acqua sono due punti qualificanti. È evidente che alcune scelte delineano un percorso da completare e altre, appena sarà possibile, dovranno essere poderosamente rifinanziate. Un esempio facile da proporre è il sostegno fiscale a favore dei contribuenti a basso reddito.

saremmo stati tutti d'accordo, avessimo avuto quelle risorse, ad aumentare di quasi 2 miliardi il beneficio a tutti. Anche i colleghi dall'opposizione, fieri oppositori di molte altre spese, oggi anche negli emendamenti propongono di rifinanziare quell'intervento. Ma è evidente che non siamo in questa situazione. Nonostante tutto ciò, la nostra maggioranza ha mantenuto la promessa, che aveva trovato formale traduzione nella legge finanziaria dello scorso anno, di ridistribuire l'extragettito fiscale ai cosiddetti incapienti. Ora la nuova finanziaria, almeno quella votata in questo ramo del Parlamento, prevede che i futuri beneficiari di un processo virtuoso di recupero

non concede al Governo - e mi avvio alla conclusione, signor Presidente - nessun alibi rispetto alle proprie responsabilità quotidiane, a partire dal rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Non sono affatto sufficienti le risorse stanziate dall'articolo 15 del disegno di legge che stiamo discutendo. Occorre quindi che nell'altro ramo del Parlamento, alla Camera, si trovino le risorse finanziarie necessarie al rinnovo dei contratti, rinnovo che va non solo a rispondere a ragioni di giustizia sociale e di equità, ma anche a ragioni di politica macroeconomica; occorre, infatti, stimolare la domanda interna. Voteremo quindi a favore di questo decreto perché riguarda complessivamente la manovra finanziaria e quindi avvia un processo di redistribuzione e di equità sociale che dovrà continuare nei prossimi anni. Noi lavoreremo con fiducia in questa direzione.

decreto-legge di cui oggi il Senato discute la terza lettura è un provvedimento su cui l'Assemblea ha già avuto modo di confrontarsi approfonditamente e - credo - con proficuo e buon esito. Si tratta di un atto di significativa rilevanza, rispetto al quale la discussione alla Camera ha introdotto poche modifiche e correttivi su cui mi soffermerò successivamente, i cui contenuti incidono già nell'esercizio finanziario 2007, e che al tempo stesso è parte costitutiva dell'insieme della manovra finanziaria che il Governo ha definito e le Camere sono chiamate ad affinare e a qualificare entro la scadenza di fine anno. Il decreto-legge, più propriamente, ha il merito di prevedere una serie di misure di spesa rese possibili dal buon andamento del gettito delle entrate erariali che ha avuto nell'anno risultati migliori rispetto alle stime previste. Va sottolineato che questa importante crescita del gettito erariale può essere considerata per larga parte di tipo strutturale, come riflesso di un allargamento della base imponibile e in quanto espressione dei risultati della lotta all'evasione e all'elusione fiscale, perché la combinazione equilibrata di controlli e sanzioni riduce la convenienza e la propensione ad evadere di molti contribuenti. Si è così potuto avviare, coerentemente con quanto disposto con la finanziaria 2007, un primo impegno di redistribuzione di risorse, con priorità alle fasce sociali più deboli, e più complessivamente la individuazione di misure necessarie e urgenti per affrontare alcuni aspetti essenziali per la politica economica, come la ripresa degli investimenti pubblici in infrastrutture e interventi di riqualificazione della spesa sociale. Certo, le misure che alla fine si indirizzano a favore dei soggetti IRPEF cosiddetti incapienti, anche per effetto della modifica introdotta nella discussione alla Camera, sono sicuramente, per i vincoli dettati dalle disponibilità di risorse, meno di quanto sarebbe desiderabile e probabilmente giusto, come aveva evidenziato anche la discussione che si era svolta in questo ramo del Parlamento. Tuttavia, resta il valore politico, oltre che sostanziale, di una misura che ha il profilo della grande attenzione a ceti e situazioni troppo spesso derubricati dalle provvidenze delle politiche fiscali e redistributive e che, se l'azione di risanamento dei conti pubblici, di rilancio dello sviluppo, di contrasto all'elusione ed evasione continuerà a produrre effetti positivi, potrà evolvere - questo è l'intento - in una misura permanente da estendere anche agli esercizi successivi a quello in corso, alla data di entrata in vigore del decreto. Così pure è significativo il primo passo che si compie con le disposizioni contenute nel decreto, relativamente, ad esempio, alla vicenda SPORTASS e non solo, verso l'unificazione degli enti previdenziali. Anche qui l'auspicio è che vi siano al più presto nuovi interventi di unificazione, per rendere più razionale e chiaro il sistema previdenziale e per consentire risparmi di spesa non indifferenti. Sotto il profilo più propriamente fiscale, poi, sono da rimarcare positivamente le semplificazioni burocratiche riguardo all'indicazione dei dati ICI nella dichiarazione dei redditi e in relazione al calcolo dell'acconto IRPEF, espressione di un rispetto verso le disposizioni recate dallo Statuto del contribuente, insieme con misure di scambio informativo tra le informazioni fiscali delle pubbliche amministrazioni utili alla strategia di contrasto dell'evasione fiscale. Così come sono importanti le disposizioni fiscali relative alla proroga della concessione del gioco Enalotto, alla trasformazione dei Monopoli di Stato in agenzia fiscale, e quelle tese alla definizione di un meccanismo più certo per la fissazione dell'addizionale comunale basata sulle aliquote dell'anno precedente e delle addizionali regionali, che possono essere modificate in senso più favorevole al contribuente, con applicazione anche al periodo di imposta al quale si riferisce la variazione.

alle aperture sul funzionamento delle conservatorie e alle disposizioni interpretative di una norma già prevista dalla finanziaria del 2007, inerente alla possibilità per i giovani, gli anziani e gli amatori, di svolgere attività

si evidenzia la natura del problema esistente nel Paese, si prende atto della difficoltà - illustrata anche dal rappresentante di Rifondazione - di utilizzare entro l'anno le risorse dei fondi dormienti e quindi si propone che vi sia un impegno del Governo ad operare nell'arco del 2008 per superare il limite dei 150 euro per ogni povero esistente nel Paese.

conti. Continuiamo ad insistere che tutta la manovra di bilancio - dal decreto "tesoretto" di luglio, a questo decreto e poi anche alla legge finanziaria - sia comunque basata su un falso in bilancio che abbiamo cercato di stigmatizzare e denunciare più volte, ma che ha visto sorda la maggioranza. Riteniamo che il conteggio per quanto concerne gli incapienti

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge che si va ad approvare in seconda lettura incide su una questione della massima rilevanza economica e sociale per il Paese, l'adozione, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica definiti con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 e con la relativa Nota di aggiornamento, di disposizioni che avviano un processo di restituzione del maggior gettito fiscale rispetto alle previsioni, dando in questo modo priorità ai soggetti incapienti ed intervenendo a sostegno della realizzazione di infrastrutture ed investimenti. Con la manovra di finanza pubblica per il 2008, attraverso importanti misure di redistribuzione sociale, il Governo dell'Unione sviluppa l'azione di politica economica e di integrazione del risanamento dei conti pubblici già preponderanti nella manovra dello scorso anno. Nella manovra per il 2007, pur essendo presenti entrambi gli elementi, il secondo era di gran lunga il più significativo, per la necessità di sanare le pendenze ereditate dalla precedente legislatura.

lotta all'evasione, recupero di base imponibile, restituzione progressiva ai contribuenti. Questi sono gli elementi di un piano che comincia ad essere attuato concretamente in sintonia con le richieste dell'Unione Europea.

che il Governo ha assunto come elemento centrale della sua politica modificando il rapporto tra fisco e contribuente, che il Governo di centro-destra aveva seriamente compromesso. L'emersione di questo nuovo extra gettito e, per un senso di giustizia, la necessità di redistribuirlo di redistribuirlo tempestivamente, sono i due elementi che hanno imposto al Governo di intervenire attraverso lo strumento della decretazioned'urgenza.

Per rendere più facile il conseguimento dell'obiettivo del 2008 il Governo, con il decreto-legge, ha anticipato alcune spese che riguardano impegni internazionali per la pace, aiuti ai Paesi in via di sviluppo per 910 milioni di euro,

Emanato dal Governo, contestualmente alla presentazione al Parlamento del disegno di legge finanziaria, il decreto-legge in fase di conversione deve ritenersi parte integrante della manovra di bilancio per il 2008,

dovuto far fronte. La *performance* dei conti pubblici per il 2007, largamente migliore delle attese, in parte da ricondursi all'extragettito tributario per il successo delle politiche di *tax compliance* messe in atto dal Governo fin dall'inizio della legislatura, ha consentito in corso d'anno di recuperare risorse aggiuntive da destinare allo sviluppo e all'equità sociale, per un importo complessivo di 14 miliardi di euro, mantenendo pressoché inalterato il programma di riduzione dell'indebitamento concordato in sede comunitaria. Se la prima manovra correttiva di 6,5 miliardi, realizzata nel luglio scorso, si connotava soprattutto per la sua portata redistributiva a favore dei soggetti socialmente più esposti (pensionati e giovani con lavori discontinui), il provvedimento attuale si caratterizza per la forte spinta agli investimenti in infrastrutture viarie su tutto il territorio nazionale. Ad essi sono destinati circa 3,4 miliardi di euro, comprensivi sia dei finanziamenti ad ANAS e ad FS per il completamento di opere stradali e ferroviarie già cantierate, sia delle nuove risorse da destinare all'ammodernamento della Salerno-Reggio Calabria e allo sviluppo della rete metropolitana nei tre più grandi conglomerati urbani nazionali nazionali (Roma, Milano e Napoli). Per altro verso, anche quest'ultima manovra espansiva, come quella di luglio, ha una significativa componente redistributiva, che incide per circa 2,2 miliardi di euro. Queste risorse sono per la maggior parte destinate ad un intervento straordinario di sostegno dei soggetti economicamente più deboli, i cosiddetti incapienti. Si tratta di un intervento senza precedenti per la sua portata: alle famiglie con redditi così bassi da non pagare imposte, che dunque non possono pienamente accedere alle agevolazioni fiscali riconosciute alle altre famiglie di lavoratori e pensionati, si riconosce un *bonus* straordinario, che viene riportato (dopo la modifica effettuata alla Camera dei deputati) a 150 euro per ciascun componente, secondo il modello dell'imposta negativa adottato con successo in altri Paesi, a partire dalla Germania. Si tratta di un intervento, innanzi tutto, nel segno dell'equità fiscale e del risarcimento sociale, che appare tuttavia significativo anche ai fini del sostegno allo sviluppo, specialmente nell'attuale congiuntura di rallentamento della crescita, consentendo di immettere nel sistema economico circa due miliardi di euro attraverso i maggiori consumi delle famiglie interessate dalle misure. Di analogo segno sociale è anche il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, già lanciato con il decreto n. che destina a tal fine 550 milioni per fare fronte all'emergenza abitativa nei Comuni ed ulteriori 150 milioni per la creazione di una società di scopo partecipata dall'Agenzia del demanio con l'obiettivo di realizzare 80.000 nuovi alloggi entro dieci anni. Queste disposizioni, unite al pacchetto di interventi fiscali sulla casa previsti dal disegno di legge finanziaria (che abbiamo già approvato in prima lettura) che prevede sgravi ICI sull'abitazione principale e misure di sostegno all'affitto per affittuari ed inquilini (più intense per i giovani), costituiscono il primo nucleo di un piano casa, con il quale il Governo intende corrispondere ad una delle più drammatiche esigenze sociali che affliggono storicamente le Città e, in particolare, i grandi centri urbani: la crisi degli alloggi. Dichiaro, dunque, il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie su questo provvedimento, che viene esaminato in seconda lettura, ritenendo quanto mai urgente convertire il decreto-legge affinché si data stabilità alle norme,

sul valore della serietà e del rigore intellettuale nella gestione della cosa pubblica. Come noto, il decreto ha rischiato di decadere a causa di un emendamento, approvato dall'opposizione e da alcuni singoli senatori collocati ai limiti della maggioranza, che raddoppiava il *bonus* per gli incapienti. Si è trattato di un emendamento che potremmo chiamare suicida, dal momento che avrebbe incrinato il complesso della sostenibilità economica del decreto. È evidente come il merito dell'emendamento fosse condivisibile. Chi non avrebbe voluto raddoppiare le risorse per le famiglie più povere del Paese? Per questo parliamo della serietà e del rigore che sono chiesti a chi ambisce a governare il Paese e, mi si permetta, a chi assume la responsabilità di rappresentare il popolo in questa autorevole sede. Strumentalità e demagogia sono comportamenti che mal si attagliano ad una democrazia matura. Oggi noi ci assumiamo la responsabilità di fare ciò che è possibile, non ciò che è auspicabile; e di spiegarlo con chiarezza ai cittadini. Alcuni hanno chiamato quei 150 euro, previsti dal decreto per cittadini incapienti, un'elemosina, come sentimmo dire in occasione dell'*una tantum* per i pensionati al minimo. Questa dichiarazione è un'offesa alla dignità di quei lavoratori e di quei pensionati che oggi vivono con poche centinaia di euro al mese e che possono trovare in quei pochi euro un attimo di sollievo. Ci piacerebbe, insomma, un Parlamento in cui vige una regola non scritta: che non si gioca per tattica parlamentare con le aspettative dei cittadini, soprattutto di quelli più bisognosi. Certamente si pone un problema vero, drammatico: la perdita di potere d'acquisto da parte dei lavoratori e dei pensionati è un dato visibile; e la crescente precarizzazione dei rapporti di lavoro, da un lato, e il costo di beni primari come la casa, dall'altro, aggravano ulteriormente la questione. Ma la soluzione a queste difficoltà, in cui versa una così larga parte della popolazione, si trova con politiche fattive, non con roboanti e inefficaci colpi di scena. L'impegno netto previsto in finanziaria affinché l'extragettito dell'anno prossimo sia destinato ai lavoratori dipendenti, le politiche per la casa previste nel decreto e nella finanziaria, la stabilizzazione dei precari: sono queste le risposte vere all'impoverimento della società cui, a causa della crescente globalizzazione, assistiamo. Serietà, rigore e giustizia sociale sono, come dimostra il complesso delle norme della sessione di bilancio, le cifre dell'azione della maggioranza. Ma noi vorremmo che serietà e rigore fossero il carattere della vita parlamentare, senza scorciatoie e infingimenti: serietà nelle spese, per qualificare la spesa pubblica; giustizia sociale nella redistribuzione nei confronti di lavoratori e pensionati; rigore nei confronti di chi pensa di poter vivere poter vivere senza partecipare alle spese dei beni pubblici, come gli evasori fiscali. Come abbiamo già avuto modo di dire in questa stessa Aula, il rigore contro l'evasione fiscale è una scelta, morale e politica, di cui si vedono oggi gli effetti; una via limpida che abbiamo intrapreso e che rivendichiamo. Non più tasse, ma che tutti paghino le tasse. Questa politica consente risposte forti e nette alle domande del Paese, dalle politiche di redistribuzione a quelle per il sapere e la conoscenza. Si pensi, ad esempio, alla scelta di aumentare di 150 milioni di euro i fondi disponibili per l'innalzamento dell'obbligo di istruzione disposto dalla legge finanziaria per il 2007, bloccando, peraltro, l'operatività della clausola di salvaguardia prevista in quella sede. Oppure, si pensi alla scelta di sbloccare i fondi per la ricerca scientifica, affidando al Ministero dell'università e della ricerca la definizione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Interventi come questi non sono rivoli, ma l'ossatura del rilancio del sistema Paese. Un maggiore investimento in sapere è infatti una premessa per costruire uno sviluppo durevole. Voglio terminare il mio intervento esprimendo una grande soddisfazione perché sono stati estesi estesi dalla Camera - e noi dobbiamo recepirlo - i benefici già riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo a quelle del dovere a causa di azioni criminose (e metto in rilievo quelle compiute dalle organizzazioni mafiose).

nel quale si è manifestata pienamente l'attività del Governo e della maggioranza, a seguito dell'approvazione della finanziaria di competenza e dei

di impiego dell'extragettito per alcune spese così come sono state identificate e discusse a tempo debito.

le proiezioni fatte) si trovano in una situazione reddituale reale inferiore rispetto all'anno scorso e agli anni precedenti. Ciò è dovuto all'aumento dei costi generali di gestione di una famiglia (per carità,

per aiutare la popolazione a basso reddito o che non ha reddito si dà un contributo, una detrazione fiscale come quella prevista nel decreto-legge

prevista dalla maggioranza di centro‑sinistra. Abbiamo preso atto che anche il senatore Fernando Rossi ha rinviato la soluzione di questo problema all'impiego di fondi dormienti nel prossimo esercizio. Prendiamo atto che in prima lettura abbiamo scherzato e un emendamento, non presentato dall'opposizione - come può succedere ed è successo - ed approvato dalla maggioranza, ma approvato da qualcuno della maggioranza che sostiene il Governo,

in termini di lotta alla povertà, cooperazione internazionale e sostegno alle istituzioni multilaterali, *in* *primis* le Nazioni Unite. Ben 40 milioni di euro vengono allocati nel Fondo italiano per le operazioni di (la cosiddetta *peace* *facility*), una struttura che risulta essere piuttosto rilevante, vista la grande difficoltà che l'Unione Africana incontra di mettere insieme truppe di *peacekeeping* che possano assolvere a compiti sempre più gravosi: basti pensare all'attuale difficoltà a costituire una forza ibrida di pace in Darfur. Si stanziano poi 130 milioni di euro per il Fondo globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi che vanno ad aggiungersi ai 260 già allocati per recuperare i ritardi nel versamento dei contributi che si erano accumulati negli anni.

una sorta di prevedibilità e sostenibilità nel lungo e medio periodo per tali contributi. Auspichiamo che il Governo voglia procedere speditamente alla costituzione di un fondo triennale che possa

100 milioni di euro sono stanziati per sostenere il Tribunale penale internazionale e il Dipartimento per le operazioni di *peacekeeping* dell'ONU. Anche in questo caso vorrei svolgere una serie di considerazioni. La prima riguarda la riforma che il segretario generale Ban Ki-moon ha attuato per le strutture di *peacekeeping*, riforma vista da alcuni in maniera abbastanza critica perché separa l'aspetto più operativo di campo da quello del *peacekeeping*, con l'obiettivo conclamato di voler aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'intervento. Questa riforma va di pari passo con un'altra che a noi preoccupa, riguardante la ristrutturazione del Dipartimento per gli affari relativi al disarmo, che viene inglobato in altra struttura: ciò rischia di rappresentare una sorta di diminuzione della rilevanza politica degli impegni per il disarmo da parte delle Nazioni Unite. giustamente e coerentemente, finanziamo le attività del Tribunale penale internazionale. Non poteva essere altrimenti, anche perché è proprio in Italia, a Roma, che il Tribunale penale internazionale venne costituito. In questo caso, si l'occasione per invitare il Governo a far sì che l'ordinamento penale internazionale interno nostro possa essere adattato alle fattispecie di reato previste dal Tribunale penale internazionale, semmai introducendone anche di nuove, qualora l'ordinamento penale italiano non lo permettesse. Così l'Italia può veramente svolgere un ruolo di grande coerenza per quanto riguarda la giustizia internazionale. Ci sono poi 410 milioni di euro di contributi alle banche e fondi di sviluppo (Banca mondiale, Banca interamericana, Banca asiatica di sviluppo). Abbiamo già avuto occasione - e vi sarà ancora domani - di discutere in Commissione di alcune questioni relative a queste banche multilaterali. La prima riguarda il tema della coerenza, ovverosia come garantire ed assicurare che gli impegni che il nostro Paese prende in queste banche, che hanno tra gli obiettivi principali quello della lotta alla povertà, siano coerenti con gli impegni che il nostro Paese assume a livello internazionale, in altre sedi, per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, e che esista quindi una trasversalità ed omogeneità di impegni per quanto concerne la cooperazione internazionale allo sviluppo. Sono banche, queste, che potrebbero rappresentare degli strumenti di lotta alla povertà ma che invece tuttora continuano a seguire un paradigma di sviluppo neoliberista, improntato alla crescita e alla liberalizzazione degli scambi commerciali. Chiediamo quindi un impegno forte del Governo italiano affinché queste istituzioni non ostino, non siano di impedimento a modelli di sviluppo autenticamente equi e fondati sui diritti fondamentali dell'ambiente e delle persone.

Signor Presidente, parlavo proprio con un cittadino che mi chiedeva se stessi al Senato: ho risposto di sì; gli ho detto anche che sarei intervenuto su questo provvedimento, recante interventi urgenti per lo sviluppo e l'equità sociale. Questo cittadino mi ha chiesto: ma che cosa intende la maggioranza per sviluppo ed equità sociale? Debbo dire di aver avuto qualche difficoltà a rappresentarglielo, perché questo provvedimento, che volete licenziare in terza lettura al Senato, sostanzialmente rappresenta tutto il contrario rispetto a quello che dovrebbe essere in un Paese normale lo sviluppo e l'equità sociale. Mi chiedo: come si può raggiungere lo sviluppo? Cercherò di spiegarlo in pochissime battute, visto il tempo piuttosto ridotto che ho a disposizione. A mio avviso lo sviluppo si raggiunge quando si creano le condizioni e i presupposti

ma non dite una cosa molto importante, cioè che mentre con una mano avete dato, alleggerendo formalmente e nominalmente il carico fiscale, con l'altra avete preso, perché avete allargato la base imponibile.

Siete stati smascherati in una maniera talmente palese che anche gli osservatori economici nazionali ed internazionali non hanno creduto alla serietà della vostra proposta. Sviluppo vuol dire anche vuol dire anche creare le condizioni per dotare il nostro Paese, che è arretrato sotto questo aspetto, di un'adeguata rete infrastrutturale. Porto solo un esempio, poiché è scomparsa dalla vostra agenda l'espressione Sud o Meridione d'Italia: in tante aree del Meridione d'Italia vi sono zone industriali dove non sono presenti le opere di urbanizzazione primaria. Non c'è acqua, non ci sono fogne, non c'è cablaggio, non c'è ADSL, non c'è linea telefonica. E voi pensate che in un Paese che deve superare diseconomie e problemi di mancato sviluppo si possano ottenere risultati positivi senza pensare per un attimo ad incrementare la dotazione infrastrutturale, non attraverso interventi a pioggia, ma attraverso interventi mirati? Non c'è nulla di tutto questo. questo. Nell'ambito di una politica che non è più solamente locale, perché la questione delle aree depresse è una questione nazionale e non solamente meridionale, non avete fatto assolutamente niente per inserire provvedimenti importanti per contrastare uno dei fattori che frena sostanzialmente lo sviluppo economico di tutto il nostro territorio, che è quello legato alla criminalità. Al contrario, avete preso in giro le forze dell'ordine e non avete creato le condizioni e i presupposti per fornire un sostegno adeguato e serio.

Non vuol dire, invece, fornire le condizioni per liberarli strutturalmente dal bisogno, creando le opportunità perché in tutte le famiglie ci possa essere un posto di lavoro, perché si possa guardare con fiducia al domani, non solamente all'obolo di fine anno? credo dovrebbero essere le condizioni per poter aprire un grande dibattito sul futuro del Paese. Magari ora sbandiererete ai quattro venti il fatto di aver creato le condizioni per dare la casa a tutti. Avete dato vita ad un programma di edilizia residenziale pubblica, ma dimenticate che le case, anche quelle legate a programmi di edilizia residenziale pubblica, debbono essere comunque pagate. Quando nelle famiglie a bassissimo reddito o addirittura prive di reddito non vi è la condizione minima per poter sopportare una sia pur ridottissima rata,

che sostanzialmente vive sugli equilibri molto spesso contrapposti tra la parte più moderata e la parte più radicale, non ha la capacità di assumere un progetto proprio per guardare con attenzione agli interessi

per guardare con fiducia al futuro. È questa la vostra gravissima colpa, che non vi addebita solo Alleanza Nazionale, non vi addebita solo chi vi parla, ma in questo momento vi addebita tutta l'opinione pubblica del nostro Paese.

avrei rinunciato volentieri a parlare su questo provvedimento, che affrontiamo dopo il passaggio alla Camera e mentre è in corso l'esame della legge finanziaria, ma sono stato stimolato stimolato dalla lettura della seconda sezione della Relazione previsionale e programmatica. Ho insistito fortemente affinché il ministro Padoa-Schioppa mandasse quella Relazione; finalmente la Relazione è arrivata e abbiamo potuto avere un quadro più nitido delle scelte pericolose e contraddittorie di questo Governo e di questa maggioranza. Non solo vengono svuotate le Tabelle A e B, e quindi tutta la programmazione legislativa; non solo si determinano risparmi virtuali sui contenimenti della spesa: avete operato una manovra espansiva netta e, circa la spesa, intervenite sui consumi intermedi ma soprattutto sulla spesa in conto capitale. Gli interventi per lo sviluppo ammontano a 13,2 miliardi, sia sull'entrata per le famiglie, con la riduzione dell'ICI e l'assegno per gli incapienti, sia sulle imprese con la razionalizzazione dell'IRES. avete preferito però una soluzione ibrida, *one off*, come si diceva una volta, che voi criticavate contro Tremonti, anziché restituire agli incapienti il dovuto che sarebbe ammontato a 1.900 euro, come ci è stato detto nell'audizione della scorsa settimana da parte dei sindacati. Vi siete fatti uno sconto di 1.750 euro, perché ne date soltanto 150, rimettete in discussione il *welfare* e l'accordo del 23 luglio. Ma i dati più interessanti di questa relazione relativo alla pressione fiscale, dove si può constatare come questo Governo abbia puntato su un più forte prelievo rispetto all'atteggiamento del Governo precedente. Un prelievo che nella componente della pressione fiscale punta sulle imposte dirette piuttosto che su quelle indirette; e le serie storiche sia del passato che del futuro ne sono una chiara rappresentazione. Se poi, signor relatore, onorevole relatore, senatore relatore, vorrà guardare la figura III.7, relativa alla spesa per interessi, potrà notare che essa cresce in misura significativa con l'avvento del Governo Prodi e crescerà progressivamente negli anni futuri, riverberandosi non solo sull'onere del costo del servizio, e dunque sul bilancio dello Stato, ma anche sul bilancio delle famiglie per i maggiori oneri sui mutui, soprattutto per quelli a tasso variabile. E voi, cosa fate? Alleviate le famiglie italiane con un intervento di 70 euro l'anno più consistenti che sarebbero necessari. Ma i risultati più interessanti dal punto di vista economico‑finanziario emergono dagli effetti della legge finanziaria e dunque dai risultati che ne derivano sul bilancio integrato.

peggioramento dei saldi finanziari e in particolare del saldo netto da finanziare che arriva a meno 33,9 nel 2008, a meno 29,7 nel 2009 e a meno 9,3 nel 2010. Non migliora il rimborso delle passività finanziarie; peggiora il saldo relativo al ricorso al mercato, passando da meno 215 Quindi, nuovo debito in valore assoluto e nuovo costo per il servizio, con tassi crescenti. Questi sono i risultati fallimentari dalla manovra. Avete applicato poi un nuovo principio per gli enti locali, quello del «più spendi, più paghi», che determinerà un aumento della tassazione locale con fattori automatici di crescita. invece i Comuni che hanno giocato d'azzardo, aiutandoli nell'estinzione anticipata dopo la scommessa (proprio una scommessa) sugli strumenti dei derivati. L'impatto espansivo della manovra si può riassumere in una lieve riduzione di entrate, una pressione fiscale che resta su livelli prossimi ai massimi storici ed un sensibile incremento delle spese nette. Per di più, gli interventi sul versante delle spese, in termini di maggiori oneri, appaiono privi di un'evidente logica complessiva che consenta di qualificarne, chiaramente, la posizione di politica economica verso la riduzione permanente del *deficit* entro i vincoli comunitari. In tal senso, l'indicatore più evidente appare nell'incapacità di frenare la crescita continua della spesa primaria a tassi superiori a quelli del PIL. La circostanza evidenzia di per sé come la correzione dei conti, pure intervenuta nel biennio 2006-2007, sia sin d'ora seriamente ipotecata dai rischi di un deterioramento per gli anni 2008-2011, nella prospettiva di eventuali peggioramenti della congiuntura economica, che si riflettano in un rallentamento della crescita delle entrate o, addirittura, in una loro diminuzione in valore assoluto, a fronte dei quali la rigidità nella crescita inerziale della spesa corrente determinerebbe il ritorno del debito pubblico su un profilo di accelerazione della crescita. In altri termini, l'elevato livello di partenza dello *stock* di debito avrebbe consigliato un approccio di politica economica più prudenziale, in modo da mettere al sicuro, per il futuro, i risultati conseguiti nel biennio 2006-2007. L'orientamento adottato invece con la manovra 2008 sembra contraddistinto da un evidente «allentamento» della morsa sui conti pubblici, al fine non taciuto di evitare uno "strozzamento" del sistema economico, dopo una risalita di 2,5 punti della pressione fiscale registrata nel biennio 2006-2007. D'altronde, è chiaro che un tale indirizzo di politica finanziaria concretizza, in ogni caso, sul piano contabile, un peggioramento di 4 decimi percentuali del *deficit* della pubblica amministrazione in rapporto al PIL, configurando una manovra di indubbio segno espansivo, su basi «finanziarie» per giunta assai precarie, essendo ancora ampi i margini di recupero sul versante della riduzione del debito pubblico e della crescita dell'avanzo primario. Difatti, nel merito delle scelte di intervento adottate, la manovra si disperde ancora una volta in una serie di microinterventi, mille rivoli, che testimoniano della difficoltà di governare la spesa corrente iscritta in bilancio. Sotto il profilo tecnico, le criticità sono per giunta aggravate dai rischi insiti nelle stesse quantificazioni delle misure introdotte, rispetto a cui, a fronte del loro valore facciale assunto nel quadro di previsione, appaiono, a ben vedere, sovrastimati gli effetti ascritti, con particolare riferimento sia ai recuperi di gettito derivanti dall'allargamento della base imponibile, che ai risparmi di spesa sul fronte della razionalizzazione degli organi politici e su quello della gestione del patrimonio immobiliare pubblico. Inoltre, è da osservare l'effetto aggiuntivo derivante dall'attuazione delle misure di tono espansivo *una tantum*, per il solo 2007, già adottate in precedenza con l'utilizzo dei cosiddetti tesoretti, per cui si creeranno (sicuramente) forti, fortissime pressioni per la loro reiterazione anche negli anni a venire, con un peggioramento del saldo di bilancio ipotizzabile in 3 decimi di punto. appare assai probabile l'eventualità che il *deficit* torni nuovamente ad essere superiore al 3 per cento nel 2009. Altro che partito del «tassa e spendi», come scriveva stamattina il presidente Dini, qui siamo oltre; è una manovra in *deficit*, in *deficit spending*, quindi da bocciare. Facciamo appello a chi ha a cuore il bene del Paese, a chi guarda dentro i conti pubblici per bocciare una manovra in *deficit*, che non può essere avallata, soprattutto per le incertezze sulla crescita che rischiano di far saltare gli obiettivi previsti, aggravando il *deficit* e, quindi, il costo del servizio. Per queste ragioni, Presidente, esprimo un giudizio fortemente critico sulla manovra complessiva.